Signor Presidente, so che spetterà alla Presidenza un ricordo più compiuto, ma questa notte è morta una grandissima personalità della storia contemporanea: l'ex presidente dello Stato di Israele, Shimon Peres, una delle grandi personalità del nostro tempo. *(Applausi)*. è stato un collaboratore di Ben Gurion, uno dei grandi fondatori dello Stato di Israele, è stato un uomo

È stato un difensore senza esitazione dello Stato di Israele e della sua esistenza, ma è stato anche un grande uomo di pace. Non a caso ha ricevuto per questo il premio Nobel e, non a caso, ha sempre lavorato per una coesistenza pacifica tra i il popolo palestinese e il popolo israeliano. Ho creduto fosse giusto, oggi, interrompere per pochi attimi i nostri lavori, per dedicare un ricordo a questa grande personalità, che è stata anche profondamente legata al nostro Paese. Ricordo che con i colleghi della 2ª Commissione (affari esteri,

edificio sul mare, che irradia pace e serenità in un'area martoriata del Medio Oriente. Signor Presidente, credo sia giusto che il Senato lo onori nei tempi e nei modi che il Presidente riterrà, ma per il momento ho ritenuto doveroso, come Presidente della Commissione affari esteri, emigrazione, prendere la parola e sottoporre a voi il ricordo di questo grande uomo e di questa grande personalità. *(Applausi)*. La Presidenza si associa alle espressioni che il Presidente della Commissione esteri ha voluto esternare nei confronti di Shimon Peres, che in tanti abbiamo avuto modo di incontrare e di apprezzare in Israele e nella sua attività internazionale. Un protagonista della storia contemporanea, per il quale credo che l'Assemblea, in attesa di altre iniziative, debba ricordarlo con un minuto di silenzio.

possono esserlo anche i grandi imprenditori e i cinema Multiplex: attori forti che in generale smuovono un inviluppo finanziario notevole

- di salvaguardare e promuovere la pluralità culturale nel settore del cinema e dell'audiovisivo, assicurando un sostegno adeguato proprio a quei soggetti deboli, che sarebbero in pericolo laddove il sostegno pubblico dovesse venire a mancare o essere ridimensionato. Da questo punto di vista, credo che il disegno di legge in esame presenti ancora notevoli criticità.

Ricordo a tutti i colleghi che inizialmente, in Commissione, stavamo discutendo un altro disegno di legge, la cui prima firmataria è la senatrice Di Giorgi, che era anche relatrice del provvedimento. Lo abbiamo cominciato a esaminare a metà del 2015, prevedendo una lunga serie di audizioni, che si sono svolte nel giro di quattro-cinque mesi e che hanno fatto sfilare davanti a noi, in Commissione, tutti gli *stakeholder* del mondo del cinema.

La vicenda del Consiglio strategico del cinema è molto interessante, da questo punto di vista. Il disegno di legge presentato dalla senatrice Di Giorgi prevedeva un Centro nazionale del cinema, che era un ente terzo molto più collegiale rispetto ad un semplice comitato ministeriale

poi essere reinserito dalla relatrice nell'articolato, cancellando la sezione cinema delle Consulte dello spettacolo presso il MIBAC. Quelli erano veramente organismi collegiali che prevedevano, tra l'altro, la rappresentanza

va a imprese che già hanno una tradizione consolidata di produzione cinematografica. Stiamo parlando delle grandi imprese e non certo delle piccole imprese indipendenti e questo è un altro *vulnus* rispetto al rappresentare la pluralità culturale di cui parlavo all'inizio.

di cultura cinematografica, ovvero le associazioni che capillarmente nel territorio mandano avanti programmi di divulgazione cinematografica attraverso le proiezioni, i dibattiti e la gestione delle piccole sale. Sono sostanzialmente quegli

per quanto modificato in Commissione da vari emendamenti, rimane del tutto insoddisfacente e - a mio parere - irricevibile nel campo delle garanzie alla pluralità culturale nel settore del cinema e dell'audiovisivo. Se si volevano garantire questi semplici valori - che definirei addirittura costituzionali - si doveva prevedere un ruolo dello Stato molto più attento a queste piccole realtà e molto meno attento alle grandi distribuzioni e alle grandi sale,

*(PD)*. Signor Presidente, credo che negli occhi di tutti noi sia rimasto quel capolavoro di Giuseppe Tornatore intitolato «Nuovo cinema Paradiso», che descriveva la storia amara,

alla sensibilità della relatrice e della Commissione, durante il lungo lavoro che è stato svolto in sede di Commissione, sono stati approvati tre emendamenti, di cui due a mia prima firma, proprio su questo tema. Sono emendamenti che vanno nella direzione di istituire una sorta di via preferenziale per il contributo per l'esercizio cinematografico in piccole sale,

Considero questo intervento come il riconoscimento di una realtà che spesso noi dimentichiamo. Nei Comuni che hanno meno di 10.000 abitanti, che rappresentano l'85 per cento dell'universo complessivo dei Comuni italiani, vive circa il 30 per cento della popolazione italiana. Ebbene, in questi anni, in questi territori si è assistito ad una devastante desertificazione, con la scomparsa di queste sale, che invece, in passato, avevano rappresentato un momento identitario di formazione culturale culturale e di idea di comunità che credo vada aiutato e salvaguardato. Ovviamente, la desertificazione delle sale è avvenuta per cambiamenti nelle abitudini e nei consumi: l'irruzione della *pay*-TV, la diffusione di Internet e anche, soprattutto negli ultimi anni, un aumento significativo dei costi per il passaggio al digitale e quindi l'adeguamento e l'innovazione tecnologica.

sottoporre all'attenzione dei partiti politici - perché la «politica» ancora non è una parolaccia e i partiti sono previsti dalla Costituzione ma anche in quella occasione il Governo ci ha presentato il dispositivo, bello e cucinato nelle segrete (ma neanche tanto segrete) stanze di Palazzo Chigi. E la stessa cosa è avvenuta con la legge sul cinema, una legge in larga misura condivisibile, che non è uno stravolgimento dei disegni di legge che erano all'attenzione dei membri della Commissione (ho anche l'orgoglio di poter dire che tra questi disegni di leggi ve ne era uno a prima firma Giro, sulle opere prime e sulle opere seconde). Tuttavia, anche in questa circostanza il Governo ha voluto imporre alla Commissione un articolato molto complesso, che abbiamo naturalmente valutato ed emendato, ma l'impianto è quello che il Governo ci ha cucinato. Ha ragione il senatore Bocchino a ricordare che noi in questi mesi, quasi un anno, abbiamo ascoltato gli operatori del settore, quindi ci siamo confrontati, grazie a un encomiabile, rigoroso

che nel 2004 partorì due provvedimenti importanti, due decreti legislativi, peraltro approvati lo stesso giorno (era un gran lavoratore Urbani, tempestivo ed efficace):

mai usciti sugli schermi cinematografici. Purtroppo, ci sono casi eclatanti, che per amor di Patria non ricorderò, perché coinvolgono registi rinomatissimi, che hanno preso, allora, miliardi di lire dopo, milioni di euro per film poco visti o mai prodotti. Questa è la realtà che avevamo alle spalle. Fortunatamente, è arrivato il professor Urbani, che sa far di conto e ha proposto di introdurre un sistema automatico o parzialmente automatico, con l'interlocuzione con una commissione di esperti di fama nazionale e internazionale che avessero un minimo di cognizione di cosa sia la produzione di film e di cosa sia il cinema.

legge, del cinema italiano, della diffusione all'estero, della vendita dell'immagine Italia nei circuiti internazionali, della logica industriale che deve soprasiedere a un settore che è primario per il benessere economico di questo Paese. Parliamoci chiaro:

per la promozione del cinema e dell'audiovisivo. Abbiamo quindi 400 milioni di euro che diamo al cinema. Benissimo, io ci sto, sono favorevole a sostenere il cinema, cinema, ma attenzione: facciamo verifiche di qualità, cerchiamo di non buttare ancora una volta, risorse, come è avvenuto in passato e per responsabilità non del centrodestra, che non ha mai avuto il controllo su nulla

che presenta la sua proposta, deve dimostrare di aver incassato con i film precedenti, cioè di fare film che destano un minimo di interesse, perché

Va bene, però attenzione: questi criteri vanno applicati con assoluta trasparenza, perché parliamo di circa 60-70 milioni di questi 400 milioni l'anno, quindi di molti soldi per le grandi produzioni.

Quindi, per quanto riguarda i contributi selettivi decide il Ministro: decide chi premiare, chi sostenere, chi favorire. E non solo: l'applicazione di tutta questa normativa è demandata ai decreti ministeriali, un antico problema, che la senatrice Di Giorgi avrebbe voluto aggirare istituendo un comitato autonomo di promozione del cinema sulla falsariga del modello francese, ma non è stato possibile.

che svolge attività di analisi, esprime pareri, organizza consultazioni, formula proposte, insomma il nulla. Io però mi fido del Governo, che è fatto da partiti politici votati dalle persone, io mi fido e mi affido al Governo e al Ministro. Ci sono dei criteri oggettivi: qualità del progetto. Quindi, affidiamoci agli esperti, perché al Ministero ci sono degli eroici, come i sovrintendenti, per i quali ho sempre avuto grande

Presidente, colleghi, dopo i numerosi rinvii è stato strumentalmente anticipato a oggi l'*iter* di esame e approvazione del disegno di legge recante la disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo. Tra l'altro, essendo un testo collegato alla manovra di finanza pubblica, avrebbe dovuto avere precedenza sugli altri provvedimenti già da prima. sono state svolte le audizioni sul testo della collega Di Giorgi, che desiderava garantire un percorso democratico per arrivare a un testo finale realmente condiviso con gli operatori del settore, come più volte ha dichiarato ella stessa ai soggetti auditi. Purtroppo, a capo del Partito Democratico c'è il signor Renzi e il Governo, ben poco democratico nei principi e nei metodi,

al fine di limitare - come sempre più spesso avviene - le prerogative del Parlamento e garantire la realizzazione di marchette richieste, dimenticando - viceversa - la definizione di documentario e fornendo un errato inquadramento delle *film* *commission*, enti che dovrebbero essere ben estranei ai giochi e alle esigenze elettorali della classe politica e usati non già per dare assistenza alle amministrazioni amministrazioni locali, bensì per garantire prioritariamente supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali, in grado di intercettare varie fonti di finanziamento

la nostra idea di cinema - come potete immaginare - si è rivelata molto differente da quella della maggioranza e soprattutto del Governo, poggiando su obiettivi alternativi e ben definiti, che sono quelli di valorizzare le professionalità e le competenze acquisite dai lavoratori appartenenti a ciascuna fase del processo di lavorazione e distribuzione della pellicola cinematografica; restituire agli investimenti pubblici sull'industria del cinema della valenza culturale e sociale, valorizzando, attraverso la promozione di un cinema di qualità, la formazione del pubblico, a partire dai giovani nelle scuole di ogni ordine e grado; garantire trasparenza e meritocrazia nell'erogazione dei contributi statali e delle agevolazioni fiscali, con un particolare occhio di riguardo a registi e prodotti cinematografici emergenti e italiani ovvero alle *start up* del settore; prevedere agevolazioni fiscali per le sale cinematografiche dei Comuni medio-piccoli, nella convinzione che nelle piccole e medie realtà territoriali le stesse sale costituiscano un elemento indispensabile di aggregazione sociale per tutte le età, come opportunità di crescita

Poco o niente è stato previsto a livello fiscale per le piccole sale cinematografiche, per le quali avevamo proposto almeno uno sgravio fiscale dignitoso del 25 per cento nei Comuni fino a 90.000 abitanti. Queste nostre proposte ben si legano alla valenza che a livello europeo viene riconosciuta alle opere audiovisive e in particolare cinematografiche, considerate come strategiche, perché rispecchiano la varietà culturale delle diverse tradizioni e le storie degli stessi Stati Stati membri. Lavorando in chiave emendativa a questo provvedimento, abbiamo perciò cercato di garantire alle professionalità italiane una tutela maggiore rispetto a quella di cui hanno potuto beneficiare fino a oggi, perché si è imposta anche in questo settore la delocalizzazione come dura legge del mercato. Molti sono i produttori che negli ultimi anni, dopo aver incassato cospicue risorse pubbliche, hanno trasferito le produzioni all'estero per risparmiare sui costi, penalizzando però molti talenti e professionalità anche storiche del nostro Paese. In merito abbiamo presentato degli emendamenti, ma il Governo ha accolto solo un ordine del giorno a mia prima firma, in cui si invita a introdurre dei meccanismi di carattere normativo per prevedere la restituzione del contributo pubblico qualora le imprese cinematografiche italiane o straniere operanti sul nostro territorio non impieghino almeno il 50 per cento di tutto il personale previsto nel progetto di produzione presentato. E auspichiamo che questo venga realmente realizzato. Un settore fino ad oggi sottovalutato, nel suo ruolo di rifinitura e di garanzia di qualità del prodotto cinematografico, è è quello della post-produzione. Anche su questo abbiamo cercato di intervenire, ma il Governo ha previsto, all'articolo 27, commi 1 e 2, per la digitalizzazione del patrimonio audiovisivo e cinematografico nazionale, solo un contributo a fondo perduto di 10 milioni di per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Noi del Movimento 5 Stelle consideriamo ormai superato il fondo perduto, un metodo di assegnazione

diversamente, che per le imprese italiane impegnate nella postproduzione ci siano l'accantonamento del fondo perduto e il collegamento dell'erogazione dei contributi pubblici sulla base di investimenti già effettuati su innovazione tecnologica, tenendo conto anche della grandezza della struttura e del grado di adeguamento della stessa alle norme di salute e sicurezza previste dalla legge; un corretto utilizzo di *software* originali; un'attenzione dimostrata per l'occupazione giovanile - aspetti legati a una seria progettualità nel breve e medio termine - e la previsione di un adeguato volume di investimenti. Esprimo soddisfazione per l'accoglimento del relativo ordine del giorno, ma speriamo che venga messo in atto. Chiederemo quindi conto di concrete realizzazioni per questi impegni. Con spirito migliorativo del testo abbiamo anche tentato di inserire l'obbligo per i produttori e distributori di dotare i film in uscita in Italia di alcuni ausili di accessibilità, come sottotitoli e audiodescrizione, per un pubblico affetto da particolari disabilità. Occorre dotare le sale cinematografiche di riceventi radio per le audiodescrizioni e occhialetti per i sottotitoli. È un progetto già attivo in Francia, in Inghilterra e nei Paesi del Nord Europa che, seppur non approvato *tout court* dalla Commissione, ha almeno imposto alla maggioranza di prevedere tra i principi fondanti della legge promuovere e favorire la più ampia fruizione del cinema anche per persone con disabilità. disabilità. Al momento, sono solo buone intenzioni, ma questa è la strada da percorrere per far nascere una nuova cultura del rispetto e della piena integrazione. Anche in questo *iter* legislativo siamo stati le sentinelle dei cittadini, con capacità di ascolto, con una visione lungimirante dell'industria del cinema, in difesa delle fasce sociali meno fortunate e dei settori

il provvedimento oggi in discussione reca misure inerenti il cinema e l'audiovisivo e contiene norme rilevanti per questi due importanti settori del nostro Paese. In Italia, il cinema è stato notoriamente oggetto, sino ad oggi, di un *corpus* legislativo disomogeneo e disorganizzato fin dai suoi primi tentativi di regolamentazione.

Il ministro Franceschini ha riconosciuto in questo senso il percorso avviato dal Partito Democratico, che ha presentato una prima proposta di legge sul tema, a prima firma della senatrice Di Giorgi, che io ho sostenuto e sottoscritto con molti altri colleghi, evidenziando il valore e la rilevanza sociale del cinema e delle sale cinematografiche e di come lo Stato si debba impegnare per la diffusione della cultura cinematografica in Italia.

legge è stato esaminato e migliorato nel corso dell'esame dei colleghi della Commissione istruzione ed è giunto infine all'esame dell'Assemblea. Come ha ricordato la relatrice Di Giorgi, che ringrazio del lavoro svolto insieme a tutta la Commissione, il provvedimento ha come obiettivo il rilancio e lo sviluppo del settore cinematografico e audiovisivo in attuazione di principi consolidati anche a livello internazionale ed europeo, a salvaguardia dei valori e delle identità culturali nella società globale e tecnologica. Oltre alle finalità e i principi, il testo contiene diverse misure di carattere finanziario, che permettono al provvedimento di avere le gambe per muoversi poi da solo. Non è quindi un investimento a costo zero: si tratta di un impiego di risorse rilevanti fatto dal Governo e dal Parlamento che va quindi sostenuto, come è stato ricordato prima anche dal senatore Fornaro. Tra le misure più interessanti, vi è innanzitutto il raddoppio delle risorse esistenti con l'istituzione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. La dotazione è aumentata a 400 milioni di euro annui (a fronte degli attuali circa 200 milioni, allocati però su diversi fondi). Circa 70 milioni di euro saranno destinati a progetti diretti prioritariamente ai giovani, alle opere prime e seconde, ai film *d'essai* e ai contenuti di qualità. Altra misura importante è il *tax credit*, che va dal 15 al 40 per cento a seconda delle tipologie e delle finalità di cui beneficerà un gruppo composito di soggetti, al fine, da una parte, di tutelare il nostro *made in Italy* e, dall'altra, di ricercare investimenti stranieri. Vi è poi un articolo importante, il 26, quel piano straordinario per le sale cinematografiche, che rappresenta un altro investimento notevole. Esso impiegherà 30 milioni di euro annui per il 2017, 2017, 2018 e 2019, altri 20 milioni per il 2020 e 10 milioni per il 2021. In totale saranno ben 120 milioni di euro di contributi a fondo perduto per cinque anni per favorire la diffusione omogenea delle sale sul territorio nazionale, con particolari agevolazioni per i centri storici e per quei Comuni con meno di 15.000 abitanti che sono veramente la maggior parte nel nostro territorio nazionale. Ulteriori contributi, 10 milioni di euro per tre anni a fondo perduto o per finanziamenti agevolati, sono stanziati per interventi di digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche da parte di imprese italiane. Infine, il disegno di legge riserva ben 12 milioni (almeno il 3 per cento del fondo) per l'educazione all'immagine, la formazione di insegnanti, l'istituzione e lo sviluppo di corsi, in accordo con il MIUR, che permetterà di creare negli anni un pubblico capace di fruire dell'offerta cinematografica in modo attento, esigente e critico. Attraverso questo provvedimento, il cinema viene finalmente considerato uno strumento di crescita, condivisione e apprendimento, fondamentale per il nostro sistema culturale. L'integrazione tra cultura e istruzione è un elemento molto importante da realizzare. Così il MIBACT e il MIUR hanno siglato un protocollo d'intesa che prevede attività di promozione del linguaggio e della cultura cinematografica e teatrale nelle scuole. L'obiettivo è incoraggiare la pratica teatrale, cinematografica, artistica e performativa nelle scuole, come esperienza formativa e creativa, sia come strumento di educazione al linguaggio artistico ed estetico e dare così seguito a quanto già stabilito all'interno del decreto la buona scuola. L'armonizzazione tra i vari Ministeri, non soltanto tra i Ministri, che dialogano tra di loro è avvenuta con l'alternanza scuola-lavoro e avviene adesso con la cultura e l'istruzione. I ministri Franceschini e Giannini hanno presentato, inoltre, due concorsi rivolti agli studenti sui temi del cinema e del teatro. un cambio di prospettiva significativo: le scuole sono andate molto spesso a teatro e al cinema, mentre oggi si porta il cinema e il teatro dentro la scuola, per riavvicinare il pubblico alla cultura. Si tratta di un ritardo a cui si sta ponendo rimedio. Voglio anche ricordare come il decreto legislativo sulla buona scuola preveda tra le materie scolastiche non solo il ritorno della storia dell'arte, ma anche l'introduzione del cinema e dell'audiovisivo, mai prese in considerazione a livello ministeriale. Anche il *bonus* cultura di 500 euro per i giovani, da spendere per teatri, cinema e musica, rappresenta un intervento importante. Detto questo, le norme contenute nel provvedimento in esame hanno tutte la finalità di razionalizzare il sistema e semplificare gli interventi di promozione e sostegno al cinema. Ritengo, quindi, opportuno un rapido esame del testo per una immediata approvazione dello stesso e il passaggio alla Camera. Faccio presente ai Gruppi che alcuni colleghi hanno rinunciato a intervenire in discussione e, quindi, la fase di votazione è imminente. È iscritto a parlare il senatore Bruni. Ne ha facoltà. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo a esaminare il disegno di legge n. 2287 per la disciplina dei settori del cinema e dell'audiovisivo. Dopo una molto "conveniente" inversione dell'ordine dei lavori, è stato infatti deciso che questo provvedimento fosse meno rischioso per la maggioranza rispetto al disegno di legge di riforma del codice di procedura penale. Rimescolate così le carte, partecipiamo ancora una volta a un gioco delle parti costruito appositamente per prendere tempo e che automaticamente sembra quasi declassare il provvedimento in esame che - come abbiamo sentito nel corso degli altri interventi che mi hanno preceduto - è invece molto importante. Sebbene non vi si trovino questioni spinose quali intercettazioni e prescrizione, chi ha partecipato al lungo *iter* di questa riforma in 7ª Commissione - come ha fatto il senatore Liuzzi per il nostro Gruppo - sa che da lungo tempo ormai si aspettava il capitolo conclusivo del provvedimento. Questo disegno di legge dovrebbe, infatti, costituire una riforma organica di un sistema che per anni è stato caratterizzato da leggi, leggine, decreti e regolamenti che hanno reso l'impianto normativo un labirinto tanto complesso quanto privo di una visione. Eppure, il cinema italiano rappresenta un'eccellenza del nostro Paese. Rappresenta lo spirito artistico e creativo che, fin dai tempi antichi, è stato prerogativa delle menti italiane. Come tale andrebbe valorizzato, protetto e esportato tenendolo sul palmo della mano. Ancora di più questo testo è figlio di un altro disegno di legge, presentato dalla collega Di Giorgi, che aveva raccolto un gran numero di consensi anche tra gli esponenti degli altri Gruppi e lo stesso senatore Liuzzi ne era stato cofirmatario. Probabilmente si trattava di una proposta migliore sotto molti punti di vista: ad esempio, prevedeva il Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive, disciplinato dettagliatamente nella sua composizione e nelle sue funzioni, per costituire un organo di autogoverno del settore. Invece, nel presente testo il Centro nazionale è stato sostituito da un generico Consiglio superiore dalla vasta attività ma dai poteri incerti, costituito da personalità di comprovata qualificazione professionale per le quali non si prevede emolumento, quindi precari o disoccupati di successo. Come spesso accade, siamo dovuti scendere a compromessi e adottare il testo proveniente dal Ministero. Fortunatamente, almeno alcune proposte emendative sono state accolte, visto che il testo del Governo non conteneva nemmeno le definizioni di «*film d'essai*» e di «sala *d'essai*», solo per citarne alcune. Non commentiamo neanche la prassi, ormai consolidata, di proporre emendamenti all'ultimo minuto, e la relatrice ‑ non me ne voglia ‑ sa bene come ciò frustri la possibilità di altri colleghi di valutare le proposte e intervenire. Tornando alle definizioni, vediamo come quella di «opera audiovisiva» comprenda pressoché tutto, ivi comprese opere dal contenuto video-ludico e soprattutto la televisione. Ci sorge spontaneo, quindi, il sospetto che la finalità ultima del progetto sia, più che altro, finanziare le *fiction*, le quali forse si vorrebbero sostituire al racconto cinematografico, che è veramente tutt'altra cosa. Un'altra parte che desta perplessità è quella relativa alle modalità di finanziamento. I contributi tratti dal Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e dell'audiovisivo sembrano essere, per l'85 per cento, quasi automatici, cioè sostanzialmente appannaggio delle imprese già posizionate nel mercato

rivolti ai film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie. In sostanza, la maggior parte delle risorse vanno alle società forti e le briciole alle produzioni indipendenti, e cioè ai film che spesso vincono i premi e si segnalano per la qualità. La percentuale attribuita alle eccellenze e ai prototipi scende poi al 10 per cento circa, essendo compresa nella quota una sequenza di voci che attengono alla promozione in Italia e all'estero. Tra le righe emerge perciò la linea del Governo: finanziamenti generosi alle grandi società di produttori e alle loro associazioni in barba all'universo degli autori e delle piccole strutture. strutture. Questi sono i contenuti principali che noi abbiamo rilevato come Gruppo dei Conservatori e Riformisti e, sulla base di ciò, esprimiamo al momento una posizione

che vedremo realizzato dopo l'esame degli emendamenti, esprimeremo una posizione più compiuta e lo farà per noi il capogruppo in Commissione, senatore Liuzzi.

ci si può "consolare con l'aglietto", come si diceva un tempo quando la nostra esperienza era più vicina al mondo dell'agricoltura. Si può, cioè, dire che nel disegno di legge è stato inserito, grazie ad alcuni emendamenti, un sostegno alle piccole sale cinematografiche, come ha fatto il senatore Fornaro, o si può dire che l'industria del cinema ha un bisogno disperato di qualche euro in più, e questo provvedimento glielo promette. ha un bisogno disperato perché - come sapete -l'industria culturale, e quella cinematografica in particolare, è confrontata con una concorrenza da tanti anni ormai assolutamente asimmetrica ed estremamente forte del prodotto americano.

la legislatura e che si possono sintetizzare in una frase: un continuo, progressivo, metodico esproprio del Parlamento da parte del Governo. Governo. Onorevoli senatori, io avevo firmato il disegno di legge a prima firma della senatrice Di Giorgi sul cinema. Non condividevo tutto di quel progetto, ma c'erano due capisaldi particolarmente importanti e promettenti, e si faceva riferimento in modo chiaro e ripetuto all'esperienza francese.

Il secondo asse portante dell'intenzione della senatrice Di Giorgi era di procedere a una metodica consultazione dei protagonisti del settore,

a sostituirsi al Parlamento e, in cambio di pochi soldi e pochi finanziamenti, a sedersi a tutti i tavoli in cui si decida qualunque cosa a proposito delle attività culturali, economiche

il disegno di legge, anch'esso di iniziativa governativa, riguardante la RAI. Vi dissi allora che quel progetto serviva sostanzialmente al Governo per sedersi al tavolo con i grandi *network* privati e regolare, di fatto, il sistema da Palazzo Chigi. Ciò è avvenuto e le stesse polemiche scomposte da parte della maggioranza nei confronti degli amministratori della RAI, che sono stati nominati dal Governo e dalla maggioranza, danno il senso del del vero obiettivo, che è una gestione *in progress* e corporativa del settore, in questo caso televisivo. Ebbene, con il cinema si vuole fare esattamente la stessa cosa: in cambio di pochi soldi si nomina un comitato, che sostanzialmente è per intero di nomina governativa, che deciderà l'allocazione dei fondi. Anche il linguaggio fa capire che il Governo intende spalleggiare e accompagnare

però, pochissimo degli autori e della cultura - che pure nel cinema è stata prodotta - e si interviene pesantemente sull'aspetto del *business*. È stato deciso di non ricorrere a una tassa di scopo, e anche questa è una decisione demagogica e sostanzialmente sbagliata. Una tassa di scopo per difendere la grande produzione culturale italiana sarebbe stata infatti apprezzata dagli italiani, i quali naturalmente non vogliono essere taglieggiati dalle tasse, ma accettano di mettere mano al portafoglio quando capiscono a cosa ciò serve. E soprattutto

il fatto che oggi ci troviamo a discutere, e poi a votare, il disegno di legge sul cinema non è neutrale. La ragione, molto semplice - va detta chiaramente in quest'Assemblea - è che il Governo non è pronto a discutere il provvedimento sulla Si è conclusa la discussione generale; si dovrebbe entrare nel merito degli emendamenti, ma il Governo non è pronto. Per chi non avesse visto, con iPad e telefonini, quello che sta succedendo, questa mattina, in un'intervista, il ministro

Senza i volenterosi del Gruppo messo su dal senatore Verdini, la maggioranza rischia. Basta una piccola botta di malumore di qualche senatore del PD, che sostiene legittimamente posizioni diverse sulla prescrizione, che la maggioranza viene meno. Per questo procediamo con l'inversione dell'ordine del giorno, e tutto ciò, come anche la scelta di sostituire il disegno di legge Di Giorgi con il provvedimento Franceschini, fa parte di un modo di governare il Paese. Noi non siamo davanti a un Parlamento che pretende troppo o che fa perdere tempo. Siamo davanti a un Governo che fa e disfa e si mette sempre al centro della scena con risultati assolutamente insoddisfacenti. legge all'esame dell'Assemblea, oggetto di lunga analisi e discussione in 7a Commissione, propone un ridisegno generale e complessivo della normativa relativa al settore del cinema e dell'audiovisivo. In origine conteneva anche norme relative allo spettacolo dal vivo, che la Commissione ha proposto di estrapolare essendosi ritenuto che questo sia un settore meritevole di altrettanta, approfondita analisi. Tale proposta di stralcio è stata apprezzata anche da varie associazioni attive nel settore che hanno comunicato la loro condivisione. Il provvedimento parte dal presupposto della concorrenza con i nuovi sistemi di comunicazione, intrattenimento intrattenimento e comunicazione - in particolare l'emittenza televisiva - che hanno creato serie difficoltà al settore, il quale ha necessità, quindi, di trarre nuova linfa da norme di maggiore attualità e, soprattutto, ha necessità di nuovi investimenti e incentivi per stimolare la competitività. È un settore, quello del cinema, che potrebbe concorrere in modo importante al rilancio dell'economia italiana, oltre a offrire nuovi stimoli di crescita culturale. Gli interventi prospettati con il disegno di legge in esame si rendono necessari a fronte del difficile contesto economico-finanziario della filiera audiovisiva nazionale. Durante i mesi scorsi la 7a Commissione, con una lunga serie di audizioni, ha consultato tutti i portatori di interessi, fra i quali le associazioni dei produttori cinematografici e audiovisivi e le principali emittenti televisive, per fotografare le criticità della situazione italiana nel contesto europeo e mondiale, e sono stati poi acquisiti i punti di vista degli operatori. I vari disegni di legge proposti sono stati, quindi, sostituiti dal collegato alla finanza pubblica del Governo, che ha fatto sintesi delle numerose proposte, ma soprattutto delle istanze e delle necessità del settore. Da qui è scaturito un testo largamente condiviso e affinato dal lavoro in Commissione, che sicuramente va nella direzione di rimuovere le criticità esistenti e dare nuovo impulso a questo settore di grande importanza nel panorama culturale italiano; settore nel quale l'Italia da sempre si è contraddistinta nel panorama internazionale. Nel provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea si riscontrano forti innovazioni negli strumenti di sostegno pubblico all'industria del settore del cinema e dell'audiovisivo, creando un fondo apposito e introducendo incentivi fiscali e contributi automatici che unificano le attuali risorse del FUS cinema e del *tax credit.*

Vari articoli del disegno di legge fissano nuove regole che, pur nella necessaria garanzia di correttezza e trasparenza, introducono aspetti semplificativi nel ricorso alla misura del *tax* *credit*. Con il Fondo cinema aumentano del 60 per cento le risorse: 150 milioni in più e introduzione di un meccanismo virtuoso di autofinanziamento alimentato direttamente dagli introiti erariali derivanti dalle attività di programmazione e trasmissione televisiva, distribuzione e proiezione cinematografica. Parte del Fondo, fino al 15 per cento, viene destinato ogni anno al sostegno di opere prime e seconde, ai giovani autori, alle *start up*, alle piccole sale. Vengono rafforzati i contributi a favore dei festival e delle rassegne di qualità. A decorrere dal 2017 poi, una percentuale fissa del gettito IRES e IVA di questi settori verrà destinata direttamente al finanziamento del cinema e dell'audiovisivo. In tal modo la filiera produttiva viene incentivata a investire e innovare e vien meno l'attuale incertezza sui fondi destinati al cinema. Il nuovo Fondo non scenderà mai sotto il limite di 400 milioni di euro annui. La nuova legge affronta poi un secondo tema altrettanto importante, che è il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e delle sale polifunzionali, introducendo un fondo di 100 milioni in tre anni per la riattivazione di sale cinematografiche chiuse e dismesse, con particolare riguardo alle sale presenti nei Comuni più piccoli, inferiori a 15.000 abitanti, e per la realizzazione di nuove sale. La costituzione del Fondo è accompagnata dalla possibilità di affidare alle Regioni, in quanto competenti in materia urbanistica, la facoltà di prevedere norme di tipo edilizio anche derogatorie rispetto agli strumenti urbanistici per favorire e incentivare gli interventi di ristrutturazione e di potenziamento delle sale. Un terzo aspetto da sottolineare è l'istituzione del registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive. La misura sostituisce l'originaria previsione di una riforma del pubblico registro previsto dalla legge sul diritto d'autore con delega legislativa e contiene misure stringenti per assicurare, attraverso il registro, controlli efficaci e la massima trasparenza nell'utilizzo nell'utilizzo delle risorse pubbliche destinate al cinema e all'audiovisivo. La norma prevede anche la libera consultazione via *internet* di tutte le informazioni relative all'assegnazione alle opere di contributi pubblici, siano essi statali o regionali, erogati da enti locali o dalle istituzioni dell'Unione europea. Viene gestita nella forma della delega al Governo la questione relativa ai rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo. Lo scopo è dettare una disciplina sistematica e unitaria, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, del rapporto di lavoro, delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo. Si tratta di un intervento assolutamente urgente per dare finalmente ai lavoratori del settore una disciplina adeguata, evitando il protrarsi di situazioni ingiuste e discriminatorie derivanti dalla mancanza di un quadro di riferimento chiaro e stabile che riconosca la dignità del settore e costituisca il presupposto per le conseguenti coperture previdenziali. sono rese necessarie, fra l'altro, anche dall'approvazione di nuove disposizioni relative al lavoro in generale.

dire basta. Già questo mi mette nella posizione di dire basta! Chiudete il Parlamento, perché tanto serve a ratificare due "consiglietti" al *Premier* su come gestire - in maniera probabilmente clientelare come sarà - dei soldi per finanziare il cinema, che è un'industria che necessiterebbe sì di finanziamenti pubblici, bisogno di diventare industria svincolata dall'assistenzialismo statale cui è legata dal 1948. Bene, già solo per questo vi dico: signori, è inutile stare qui a discutere.

non c'è questo piano e non perché non siete capaci ma perché non lo volete fare, perché con questo sistema si mantengono le clientele. Cosa credete, che non abbia visto com'è finito il cinema, ad esempio, a Torino quando avete messo

è un sistema in cui, alla fine, si concentra tutto nelle mani di una persona che deciderà chi favorire tra i suoi amici. Di sicuro non ci saranno nuovi registi emergenti se continuate così. Si continueranno a finanziare film, a volte buoni ma spesso scadenti, di persone a cui un produttore non non farebbe mai fare un film perché non portano a casa niente. Perché poi il cinema, lo ripeto, è un'industria quindi va bene valorizzare il prodotto culturale ma deve marciare da sola

*(PD)*. Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il cinematografo talvolta è arte ma è sempre industria.

rientrano, secondo il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tra le eccezioni culturali. Il cinema e l'audiovisivo, infatti, sono considerati fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di aggregazione sociale in grado di rafforzare e veicolare l'identità di una comunità. A distanza di alcune settimane dall'incardinamento del provvedimento in esame va annoverata la proposta del ministro Franceschini che, in accordo con le associazioni di categoria ANEM, ANICA e ANEC, permette l'accesso alle sale cinematografiche aderenti al progetto con biglietto calmierato a soli due euro nel secondo mercoledì del mese a partire di settembre. Quindi si è già già avuta la prima edizione. «Cinema2day», che richiama le politiche culturali di incentivazione delle visite musei e i 500 euro disponibili per i diciottenni che sono già stati qui richiamati, ha già ottenuto oltre 3.000 adesioni. Sicuramente la familiarità con il linguaggio cinematografico è maggiore rispetto ad altri settori delle arti performative, come ci dicono anche le statistiche riferite alle fasce più giovani. Buona l'idea di rafforzare la fidelizzazione al grande schermo; giusto ricominciare a uscire e ridare vita a una fruizione collettiva; significativo incentivare il vivere e il condividere le emozioni; fondamentale ripopolare le sale di prossimità e, di conseguenza, dare vita ai quartieri più o meno periferici delle nostre realtà urbane, compresi i piccoli Comuni dove il cinema, laddove ha resistito, è spesso il solo presidio culturale, come si è già detto in questa discussione generale Il Governo ha dunque deciso di investire a tutto tondo in questo ambito, incrementando del 60 per ritenendolo parte essenziale della nostra cultura, capace di veicolare la nostra identità nazionale. Una storia di grande bellezza tra le tante del nostro ingegno creativo. Lo fa con una norma che interviene in modo sistemico sul cinema e sull'audiovisivo, intervenendo su tutta la filiera, dagli autori ai gestori delle sale, attribuendo le competenze a Stato e Regioni, rafforzando l'esperienza delle *film commission,* istituendo il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, e puntando sulla qualità, sull'innovazione e sulla internazionalizzazione Sappiamo che la volontà e la proposta del Governo, con questo collegato alla manovra di bilancio 2015-2017, si sono incrociate e positivamente contaminate con il disegno di legge n. 1835 di iniziativa parlamentare, di cui sono convinta firmataria. Il testo finale, ora in discussione, è il frutto

grazie al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, si ridisegna il FUS cinema e il *tax credit*. Il fondo è alimentato sul modello francese e abbiamo già ricordato più volte come opererà: a decorrere dal 2017 una percentuale del gettito IRES e IVA di questi settori,

piccole sale ubicate in paesi inferiori ai 15.000 abitanti. Si istituisce poi un fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; vengono rafforzati i contributi a favore dei *festival* e delle rassegne di qualità; è previsto un piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

precedentemente, mi riferisco all'articolo 9, che entra nel merito degli aspetti formativi sia riferiti alle specifiche professionalità coinvolte sia facendo sponda alla legge di riforma della scuola nella valorizzazione di linguaggi artistici e multimediali anche tecnologicamente avanzati, per la formazione di cittadini produttori e fruitori critici di cultura. Si parla di minimo 12 milioni che, all'anno, vengono previsto dall'articolo 25, cioè il 3 per cento Sappiamo che sono già all'attivo proficue progettualità e sappiamo che con i tre decreti legislativi previsti dalla legge n. 107 del 2013, e in particolare quello sulla cultura umanistica e di valorizzazione delle arti, si intende potenziare l'offerta formativa su questi linguaggi performativi multimediali. Diciamo che questi provvedimenti si tengono. La normativa affronta anche il tema dello stato dei contenitori, cioè degli edifici che sono interessati da diverse misure volte alla ristrutturazione, anche mediante ampliamenti volumetrici in deroga agli strumenti urbanistici

fino al 2021 e anche in questo caso i Comuni con meno di 15.000 abitanti hanno una quota parte del fondo destinata a loro. Viene riconosciuto un grande valore anche alle sale storiche e di particolare interesse culturale:

tanto degli imprenditori del settore cinematografico e audiovisivo, quanto dei principali agenti educativi (di questo non si è parlato, mi sembra di non avere sentito nessuno), tra i quali in primo luogo la famiglia, e sostituendo le procedure attualmente vigenti con un meccanismo di responsabilizzazione degli operatori e di attenta vigilanza delle istituzioni orientata all'effettiva tutela dei minori. Un ultimo rilievo va riservato alla decisione (che ritengo corretta) di proporre all'Assemblea lo stralcio dell'articolo 34 relativo al nuovo codice dello spettacolo dal vivo. Sarà questa un'occasione fondamentale per valorizzare un settore che aspetta da tempo nuove misure normative; un settore cui va attribuito un alto valore umanistico che deve incrociare - come ho detto - le politiche formative, di cui la nostra società ha estremo bisogno.

con una patologica impossibilità di programmazione, necessita di misure di semplificazione burocratica, fatica a far emergere le proprie risorse sul piano internazionale e altro ancora. Riprenderemo immediatamente i lavori di ascolto dei diversi portatori di interesse per amplificare e dare maggiore attenzione, anche in termini di sostegno, alle misure contenute in quella delega al Governo, anch'essa prevista come collegato alla manovra finanziaria. La 7a Commissione del Senato ha già lavorato per indagare sullo stato dell'arte (quanto mai corretta questa definizione) anche per quanto riguarda il *welfare* dei lavoratori del settore. Lo ha fatto nello specifico per la musica, ma naturalmente si affronterà il problema dello spettacolo in generale. Sappiamo quanto sia complesso il lavoro che ci attende, ma lo affronteremo con lo spirito che ha animato in nostro percorso rivolto al cinema e all'audiovisivo. Anzi, l'esito di questo collegato, che seguiremo con attenzione anche nelle fasi dei decreti legislativi con i pareri che

la nostra collettività, perché è in grado di creare contesti facilitanti le relazioni, l'inclusività, la multiculturalità, l'ascolto e la libera creatività, segni ed emozioni che legano performanti e pubblico. Insomma, per dirla con Tonino Guerra, grande artista, poeta e sceneggiatore, se noi imparassimo a parlare, gli animali ci capirebbero meglio. Le immagini sullo schermo vivono perché sono guardate.

questo nostro provvedimento hanno potuto notare quanti contenuti ci sono e come davvero si possa parlare di una riforma che è qui in solido. Abbiamo una riforma del cinema che mette ordine

a votare sia un po' ingiusto. Abbiamo infatti dato molta, ma molta attenzione ai giovani; abbiamo messo in campo finanziamenti per le opere difficili; abbiamo valorizzato i film e le sale *d'essai*. Abbiamo fatto

davvero si possa essere soddisfatti. Certamente lo sono io. Ringrazio i colleghi e ringrazio in particolare i colleghi delle opposizioni, che in Commissione hanno fatto un lavoro molto serio e dei quali sono stati accolti molti emendamenti nel testo

ribadire il lavoro di collaborazione tra Governo e Commissione e il miglioramento che è stato apportato al testo, anche grazie al lavoro svolto in Commissione, recependo proposte emendative di varie forze politiche. Mi riservo di intervenire nel corso del successivo dibattito che si svilupperà in Assemblea sui vari emendamenti

il film documentario. In Commissione pareva che fosse impossibile trovare una definizione di film documentario. Infatti l'emendamento è stato respinto perché nessuna delle definizioni sulle quali ci eravamo confrontati, neanche quella che alla fine avevamo proposto come Movimento 5 Stelle, pareva essere

che a noi non piace del tutto. Soprattutto ci chiediamo come mai, quando il Movimento 5 Stelle ha avanzato questa proposta, la relatrice, i funzionari dell'ufficio legislativo del Ministero e il Governo hanno sostenuto che fosse indefinibile un'opera documentaria; e poi sbuca l'emendamento della relatrice. Pare

definire con maggiore precisione le opere filmiche, ci pareva sensato introdurre anche questo tipo di definizione.

definizione di *start up*. Se, poi, la definizione da noi proposta non dovesse del tutto piacere alla relatrice e al Governo, quantomeno chiedo che possano accettare la trasformazione del nostro emendamento in un ordine del giorno per farsi carico di tale

«film a prevalente finalità culturale comprendenti anche i film di ricerca e sperimentazione», che non sono gli unici. Anche in questo caso vorremmo indirizzare a un'integrazione che consideri il tema più ampiamente.

senatrice Montevecchi, lei sa che abbiamo lavorato moltissimo sulla definizione di documentario e vi abbiamo dedicato alcune sedute, perché era difficilissimo. Nemmeno in Europa è stata trovata La formula che lei propone è molto discorsiva. Essendo tutti d'accordo sul fatto che il documentario è una forma espressiva,

noi, a un testo normativo. Quindi, ho pensato di introdurre la mia definizione, facendo in questi ultimi giorni che comunque raccoglie ciò che c'era nel vostro testo, ma espresso con una modalità che per me è di maggiore soddisfazione. Ho spiegato in questo modo l'arcano.

Esprimo parere conforme a quelli espressi dalla relatrice, facendo notare come per l'ordine del giorno G2.300,

che addirittura è stata indicata in maniera precisa cos'è un'opera prima, un'opera seconda, un'opera di animazione, un'opera audiovisiva di nazionalità italiana e così via, quindi c'è stata una precisazione, non capisco non capisco assolutamente perché non venga fatta una distinzione tra il lungometraggio e il cortometraggio. Questo è fondamentale, perché la tecnica

ci sono addirittura anche dei *festival* specifici per l'uno e per l'altro. Quindi non riesco veramente a capire - e non l'abbiamo ancora capito - perché il Governo non accetti

che è una definizione innovativa che non mi sento di accogliere. Per quanto riguarda la seconda parte sono favorevole. Il parere dunque sarebbe favorevole

alla luce delle modifiche intervenute sul testo e in considerazione delle riflessioni del senatore Conte, anche considerando lo stralcio dello spettacolo - qui si parla di sale teatrali il Governo si rimette all'Assemblea. Per il resto degli emendamenti, i pareri del Governo sono conformi a quelli della relatrice. Per quanto riguarda gli ordini del giorno,

il Senato approvava

credo che su questo aspetto sia il Governo a dover dare una risposta. Io manterrei il mio riteniamo di non accogliere l'ordine giorno con questa formulazione perché si andrebbe a creare una nuova qualificazione giuridica, quella dei presidi culturali, che riteniamo ultronea rispetto al testo della legge.

la relatrice ha dato parere contrario, che qui si chiedeva un coinvolgimento specifico e qualificante degli effettivi detentori dei saperi professionali del settore. Se dobbiamo fare l'educazione al cinema e all'audiovisivo all'interno delle scuole, non possiamo continuare a considerare i docenti come tuttologi di ogni cosa

in questo caso non accetto di trasformare un impegno in una valutazione dell'opportunità. Le vicende di Cinecittà sono note a tutti e si trascinano da tempo. Il Governo avrebbe già dovuto valutare abbondantemente quanto quanto sta accadendo a Cinecittà, e dovrebbe impegnarsi, una volta per tutte, a porre fine a una situazione veramente vergognosa per un luogo che tanto ci ha dato nel mondo, a livello di immagine e di tanto Se il Governo non ci vuol mettere mano, la ragione ha un nome e cognome ben preciso, che è già stato fatto dal mio collega Airola.

più trasparente e pubblico il lavoro del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo. Crediamo infatti che un organismo come questo

di questo che si propone di essere un organismo importante con un ruolo fondamentale per il settore del cinema, le informazioni siano trasparenti, pubbliche e accessibili. Con l'emendamento invece, ci siamo posti la preoccupazione di dare una cadenza programmata

chiedo all'Assemblea di valutare l'opportunità di inserire quanto previsto da questo emendamento e, quindi, di votare favorevolmente. L'emendamento 9-*bis*.307 non prevede altro che

al comma 3. Al comma 3, lettera *b)*, laddove si incentiva la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese, si chiede di inserire «legata al territorio». Questo è importante, perché noi incentiviamo la nascita di nuove imprese, però

**Il Senato non approva**.

desidero ricordare in quest'Aula la figura del senatore Riccardo Triglia, che è mancato proprio nello stesso giorno in cui è mancato il presidente Ciampi, del quale il senatore Triglia è stato sottosegretario quando Ciampi era Presidente del Consiglio. Riccardo Triglia è stato senatore della Repubblica dal 1979 al 1994...

Triglia è stato Sottosegretario alle finanze nel Governo Ciampi, è stato a lungo presidente nazionale dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia, presidente dell'Union of local authorities, componente della Commissione bicamerale per le riforme guidata da Aldo Bozzi. Questi sono solo alcuni degli incarichi molto rilevanti che, a livello nazionale ed europeo, il senatore Triglia ha ricoperto nel corso della sua intensa vita politica. Riccardo Triglia era nato a Casale Monferrato nel 1937 e durante tutto il corso della sua vita politica è rimasto coerente all'ispirazione di quella sinistra democristiana che ha avuto in Piemonte, con figure come Donat Cattin e Bodrato, un punto di forza e di riferimento assoluto, anche a livello nazionale, connotato dalla peculiare ed originale attenzione alla questione sociale, ai temi legati all'esperienza della fabbrica e del sindacalismo di matrice cattolica. Di questo *milieu* politico e culturale Riccardo Triglia è stato esponente di spicco, svolgendo nel contempo un prezioso collegamento tra il livello nazionale e quello locale, contribuendo a formare una nuova classe dirigente,

della Eternit, dell'amianto a Casale Monferrato, che proprio da quel nucleo politico di amministratori locali ha avuto il primo ed importante spunto. Riccardo Triglia è stato al tempo stesso, caparbiamente, un uomo del territorio e delle comunità locali,

nella quale si possono leggere ora tanto l'ostinata difesa del ruolo e delle funzioni del governo locale, quanto la preveggente intuizione, particolarmente significativa in una realtà connotata dall'intensa frammentazione amministrativa, che la difesa del ruolo e delle funzioni del governo locale può realizzarsi solo nello svolgere quelle funzioni in maniera associata. Sappiamo quanto questo tema

Nella seconda metà degli anni Ottanta, in alcuni centri non secondari dell'alessandrino, e tra questi Casale Monferrato, maturò un significativo incontro, proprio sul terreno del governo locale, tra il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana

Il sindaco sa bene che non può farlo: un amministratore pubblico non può rifiutarsi di applicare una legge dello Stato approvata democraticamente dal Parlamento. Si configura un'omissione d'atti d'ufficio, reato punibile con la reclusione da sei mesi a due anni. Se non vuole applicare le leggi italiane, può dimettersi da sindaco: gli diamo subito un consiglio. Allora, se lo sa, e non vuole delegare, che cosa accade? Ha bisogno di dimostrare a qualcuno che non vuole farlo? Oppure è solo alla ricerca di pubblicità e notorietà? Ovviamente è già su tutti i giornali ed è per questo che non lo cito: non ricordo il suo nome perché non voglio portare neppure una goccia al suo mulino. Purtroppo, però, questo non è un caso isolato. Ma i contrari devono farsene una ragione: la legge c'è ed è compito della magistratura farla rispettare. È evidente che la coppia può rivolgersi altrove, in un Comune limitrofo in cui il sindaco è più disponibile, ma tutte le lotte per i diritti hanno ottenuto questo? La legge sulle unioni civili dà certezza ai diritti, non è una legge possibilista legata alla buona volontà di qualcuno che la applichi. È paradossale: pensate se domani mattina un sindaco decidesse di non dare la cittadinanza a una persona che ha i requisiti per richiederla

I numeri sono piccoli e, tra l'altro, identificano sempre un'Italia a due velocità: fino a ora le unioni civili sono state ventisei a Milano, diciannove a Torino, nove a Roma e una sola a Napoli. I numeri sono piccoli, perché ancora molti non hanno il coraggio di utilizzare fino in fondo il loro diritto. Abbiamo fatto una legge che dà diritti, che aiuta lo sviluppo di una cultura dei diritti e della tolleranza ma, certo, il sindaco in questione dimostra che ancora molta strada resta da fare. Anzi, sindaci come questi ci fanno fare passi indietro, perché alcune coppie spaventate dalla possibile pubblicità che può essere data alla loro unione ci pensano due volte prima di chiedere un loro diritto. Molte coppie «omo» vorrebbero essere trattate esattamente come le coppie «etero», che magari vogliono sposarsi nella riservatezza, nella semplicità. Molte coppie «etero» convivono e non hanno nessuna intenzione di sposarsi e, allo stesso modo, non tutte le coppie «omo» sentono il bisogno di unirsi civilmente. La legge norma anche i diritti delle convivenze questa è un'altra parte della legge, molto importante, alla quale non è stato dato sufficiente risalto perché è stata travolta dalla grande pubblicità data alle unioni civili. però, questo sindaco che questa, come le altre coppie, non sarà lasciata sola nel rivendicare un diritto che lui non può negare. Se ne faccia una ragione: è un sindaco di un Comune italiano e, come tale, non ha potere di legiferare, ma solo di applicare le leggi. Se non vuole fare ciò che la legge gli impone, si dimetta. Noi sicuramente non sentiremo la sua mancanza.

abbiamo a che fare con la recente decisione della RAI di chiudere la trasmissione televisiva chiamata «Ambiente Italia»: una trasmissione storica che ha più di Decide di punto in bianco di chiuderla e di negare a tutti gli italiani un prezioso patrimonio d'informazione ambientale. È una decisione che, da un lato, non sorprende; dall'altro, sorprende che la decisione nemmeno tenga conto dello *share* il dio *share* - visto che la trasmissione ha buoni ascolti. Quindi, sembra evidente - tristemente, dolorosamente evidente - che la RAI voglia ridimensionare, sia per durata sia per collocazione, una parte degli spazi d'informazione dedicata all'approfondimento sul patrimonio ambientale e culturale del nostro Paese: due cose che sono e saranno sempre più importanti. Questo, tra l'altro, senza prevedere un'alternativa davvero efficace e valida. A riprova A riprova di questa dichiarazione è il fatto che la scomparsa di «Ambiente Italia» segue la recentissima decisione su «Scala Mercalli», un'altra trasmissione molto autorevole dedicata sempre ai temi del clima, dell'ambiente e delle energie rinnovabili:

Tutto questo avviene proprio mentre l'Italia, dopo gli Stati Uniti e la Cina, si prepara a ratificare gli accordi di Parigi sul clima del dicembre 2015, i famosi COP21. Tutto questo avviene mentre la sensibilità dell'opinione pubblica verso queste tematiche è sempre più forte, sia al livello nazionale, sia al livello internazionale. Papa Francesco si appella oramai quasi quotidianamente al rispetto dell'ambiente e di chi lo abita, ed è fortemente significativo che a parlare chiaro e tondo di questi temi debba essere un personaggio religioso, visto che la politica non ne parla in maniera così chiara e precisa. Per queste ragioni chiediamo al Governo di pronunciarsi sulla vicenda, considerando peraltro che, in base al contratto di servizio, rientra tra gli obblighi della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo la predisposizione di programmi di contenuto culturale, anche con riferimento alle tematiche ambientali.